ha istituito «la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» e che per la carta è stato stabilito un «importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico»; anno scolastico»; nel decorso anno scolastico 2015/2016 detto importo di 500 euro della carta è stato corrisposto ai docenti di ruolo, come prima erogazione, con accredito sullo stipendio di ottobre 2015, le spese sostenute dal primo settembre 2015 completamente ricomprese nella rendicontazione di fine anno scolastico. Pertanto il primo problema è che questa rendicontazione è rimasta sostanzialmente virtuale in quanto fatta con criteri non ancorati, nella sostanza, alle procedure elettroniche promesse attraverso un apposito decreto. Infatti, il comma 122 ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica di cui al comma 121. 121. Il problema è che dal primo passaggio al secondo sono trascorsi di fatto più di diciotto mesi. Sarebbe quindi nelle intenzioni degli interpellanti poter comprendere, attraverso un'attività di monitoraggio del Ministero, cosa è successo nel frattempo, come sono stati impiegati questi soldi, con che tipo di risposta da parte dei docenti e, soprattutto, quali sono in comparazione i numeri che caratterizzano il primo passaggio rispetto al secondo che, prevedendo l'utilizzo di procedure elettroniche, evidentemente pone il problema di un'alfabetizzazione digitale del personale docente che deve far fronte in questo modo ai propri bisogni.

che ci impone di chiedere se non intenda il Ministero provvedere all'individuazione di modalità transitorie atte a consentire nell'anno scolastico 2016-2017, a quanti hanno anticipato spese certificabili rientranti negli acquisti consentiti dal citato comma 121, il recupero delle relative somme al fine di ripristinare l'elementare certezza del diritto e la fiducia nelle istituzioni, nonché sostenere davvero l'iniziativa libera dei docenti di curare la propria formazione. PRESIDENTE. Il rappresentante

Signora Presidente, l'atto di sindacato ispettivo in discussione riguarda le modalità di attivazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Giova ricordare, in primo luogo, che in data primo dicembre 2016 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha sostituito il precedente con il quale, in via transitoria, si sono disciplinate le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per il precedente anno scolastico 2015-2016. Per assicurare l'immediata corresponsione dell'importo nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2015-2016, difatti, il suddetto importo è stato assegnato ai docenti di ruolo mediante ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria per il 2010, ossia mediante il cosiddetto cedolino unico. L'utilizzo del cedolino unico è stata una misura transitoria, come ribadito dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, la quale ha precisato che la soluzione adottata per l'anno 2015 è da considerarsi «provvisoria e straordinaria» e che non vi è disponibilità a proseguire con la gestione di NoiPA per l'anno 2016-2017. Relativamente, infatti, all'anno scolastico 2016-2017, è possibile, a partire dal 30 novembre 2016, attraverso l'applicazione *web* Carta del docente, disponibile all'indirizzo cartadeldocente.istruzione.it, effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni ed i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma. Ogni docente, mediante l'applicazione, può generare direttamente buoni elettronici di spesa con codice identificativo associati ad un acquisto di beni servizi consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dietro esibizione del precitato buono. Con riferimento, come evidenziato dall'onorevole interpellante, alle somme già spese per formazione dei docenti dal 1° settembre al 30 novembre 2016 e relative all'anno scolastico 2016-2017, Consiglio dei ministri 28 novembre 2016, è stato stabilito che le stesse sono registrate dal docente in piattaforma (così da consentire la relativa decurtazione dal borsellino elettronico della corrispondente somma) e, tramite l'applicazione medesima, comunicate al MIUR, che provvederà, previa rendicontazione delle istituzioni scolastiche, a fornire apposito finanziamento finanziamento alle istituzioni scolastiche di servizio dei docenti, le quali provvedono a loro volta all'erogazione ai diretti interessati. Infatti, con nota protocollo n. 5314 del 10 marzo 2017 sono state fornite le istruzioni operative alle istituzioni scolastiche per la suddetta rendicontazione delle somme spese nel periodo 1° settembre 2016 - 30 novembre 2016 e relative all'anno scolastico 2016-2017. Dal 19 aprile del corrente anno questa amministrazione, ai fini della gestione delle autodichiarazioni presentate dai docenti per il citato periodo, ha abilitato tutte le istituzioni scolastiche ad operare sul portale SIDI. Con avviso pubblicato nel portale SIDI in data 28 giugno 2017, il termine per dette operazioni è stato prorogato al 15 luglio. La società CONSAP erogherà gli importi relativi alle spese validate e ritenute ammissibili direttamente alle istituzioni scolastiche, che provvederanno a rimborsare i docenti che hanno presentato l'istanza di rimborso. Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa alcuna forma di discontinuità nell'erogazione del beneficio di cui al citato comma 121 della legge n. 107, che piuttosto continua ad essere garantito solo con modalità diverse, ma tutte ugualmente efficaci.

corredato da un contenuto di carattere amministrativo volto al monitoraggio dell'attività amministrativa collegata all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fa riferimento alla legge n. 107 del 2015, ma è anche un atto che ha un significato politico. Credo che, nel dichiararmi parzialmente soddisfatto e lodando la struttura del Ministero e il Sottosegretario che in Aula ha voluto rendere noti alcuni dati chiave, non posso fare a meno di notare che c'è una data che dà il senso politico di questa vicenda,

una data pericolosamente vicina al 4 dicembre 2016, e che forse doveva far significare che arrivava in tempo per poter mandare messaggi di contenuto politico che non solo non sono stati intesi, ma sono stati fortemente contraddetti. Lo dico perché l'incuria dei primi diciotto mesi è un tutt'uno con questo senso alternato di fare riferimento a un importante settore della vita pubblica del nostro Paese, la scuola, che, ripetendomi ripetendomi nelle espressioni che hanno descritto la mia interrogazione, ha bisogno di certezza del diritto e di reale cura per il destino di una generazione.

l'onorevole interrogante, prendendo spunto dalla situazione in cui si sarebbero trovati alcuni ragazzi con disabilità frequentanti le scuole del Comune di Vigevano, i quali avrebbero rischiato di rimanere dal 2 marzo scorso privi di assistenti alla persona, richiama la necessità di chiarire le competenze in materia di prestazione dei servizi di assistenza, così come richiesto dall'ordine del giorno a sua prima firma approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno». In primo luogo corre l'obbligo di evidenziare come questo Ministero tenga in grande considerazione la problematica segnalata dall'onorevole interrogante. Alle diverse iniziative attuate nel tempo si è, da ultimo, aggiunto il decreto legislativo n. 66 del 2017, con cui è stata esercitata la delega conferita al Governo con l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge n. 107 del 2015, per riordinare la materia relativa all'inclusione. Il citato decreto legislativo, all'articolo 3, individua e riordina le prestazioni e le competenze per l'attuazione dell'inclusione scolastica fra Stato, Regioni ed enti locali. Principale novità del testo è che, per la prima volta, nell'ambito della definizione dell'organico del personale ATA, si terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del genere di ciascuno studente. In particolare, secondo quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 3, gli enti locali, nel rispetto riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992; i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilito dall'articolo 26

112 del 1998; l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1,

Venendo ora al caso specifico segnalato dall'onorevole interrogante, relativo al Comune di Vigevano, si riferiscono le informazioni acquisite dal competente ufficio scolastico regionale (USR) per la Lombardia, che ha rappresentato a questo Ministero che quanto esposto nell'articolo di stampa su «La Provincia Pavese» del 2 marzo 2017, pur corrispondente al vero nella quantificazione numerica della distribuzione degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Vigevano, ad oggi risulta superato. Difatti, con lettera inviata in data 3 marzo 2017 ai sindaci dei Comuni ubicati nel territorio della provincia e agli uffici di piano, a firma del presidente e del vice presidente e consigliere delegato all'istruzione e alla coesione sociale, l'amministrazione provinciale di Pavia ha comunicato che la Regione Lombardia, con nota del 2 marzo 2017, ha espresso la volontà di assicurare il completamento dell'anno scolastico in corso, provvedendo a trasferire alla Provincia di Pavia l'importo spettante per il periodo gennaio-luglio 2017. Con la medesima nota, l'assessore regionale all'economia, alla crescita e alla semplificazione ha segnalato che la competenza e i relativi oneri delle prestazioni in questione saranno a carico della Regione Lombardia dal mese di agosto 2017. Conseguentemente, ad oggi, la problematica segnalata risulta risolta: i finanziamenti e la continuità del servizio sono garantiti e, pertanto, tutti i ragazzi con disabilità residenti a Vigevano

saranno sicuramente noti. Oltre questo chiarimento interpretativo che avevo chiesto sul riparto delle competenze, voglio ricordare che effettivamente la Regione Lombardia, anche con le recenti linee guida approvate dalla Giunta regionale con uno stanziamento di 8,5 milioni di euro, si prende in carico

troviamo in qualsiasi realtà della nostra Nazione ma, in questo caso, sulle persone disabili non si può in nessuno modo risparmiare. Tornando alla Regione Lombardia, mi fanno piacere le parole sulla risoluzione di questo caso specifico di Vigevano. Comunque, tornando alle linee guida che ho citato prima, questi 8,5 milioni di euro che la Regione darà per i servizi al trasporto e all'assistenza dei giovani disabili porteranno a una riduzione delle ore di assistenza che, per ogni ragazzo, sarà tra le cinque e le dieci ore (attualmente